con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente», della seduta pomeridiana di ieri è iniziato l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti all'articolo 7

ripresa. Il relatore mi fa presente che per concludere i lavori ha bisogno ancora di un quarto d'ora.

legislazione, un organismo *ad hoc,* quindi infarcire la legislazione di norme manifesto mi sembra oggettivamente eccessivo. In secondo luogo, è un dovere della pubblica amministrazione usare con oculatezza le risorse. Ricorrere ad una disposizione normativa che invita a fare ciò che la pubblica amministrazione deve fare, ossia usare con oculatezza le risorse, mi sembra, di nuovo, eccessivo. Semmai penalizziamo i comportamenti sbagliati.

sia molto difficile sottoscrivere una disposizione che invita altri a fare cose che noi per primi non facciamo. Basta fare un rapido giro in qualunque Commissione, ancor più nel corso della sessione di bilancio, per trovare quotidianamente almeno una sequoia di documenti inutilizzabili ed inutilizzati

8.200 è finalizzato ad individuare risorse per l'evento alluvionale che ha colpito la provincia di Vibo Valentia il 3 luglio 2006,

al 23 gennaio 2009, di fatto riconoscendo una situazione di disagio sul territorio. Ancora ci sono una serie di problemi irrisolti: molte famiglie sono senza abitazione, alcuni insediamenti turistici risultano chiusi, il territorio è ancora a rischio, non essendo stato predisposto un piano per la sua messa in sicurezza. L'emendamento da

Gli ultimi eventi alluvionali del dicembre scorso e quelli successivi di gennaio hanno costretto il Governo a dichiarare lo stato di emergenza su tutto il territorio nazionale. Successivamente, essendo stato l'evento

il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza per la sola Regione Calabria. Ci sono danni ingenti su tutto il territorio che va dalla Provincia di Reggio Calabria fino a quella di Cosenza, attraversando ininterrottamente tutta la Calabria. tenga conto che neppure i morti sono stati salvati da questo evento, perché un paesino della Provincia di Cosenza, Fagnano Castello, ha avuto anche il cimitero distrutto dagli eventi alluvionali.

che nella finanziaria 2009 è stato inopinatamente azzerato. Esso aveva una dotazione, per il 2008, di 138 milioni,

che se non si interviene per prevenire i danni possibili in caso di eventi eccezionali e per mettere a disposizione del sistema della protezione civile

quando piove un po' più del normale, i danni e le vittime sono sempre drammaticamente elevati. Ripeto, penso che sia uno scandalo e una vergogna che questo Governo

che rifiuti, si ostini con la sua maggioranza a non riconoscere un dato di fatto: la fragilità del territorio in Italia è un grande problema nazionale, un problema di sicurezza dei cittadini, un problema sociale ed anche economico, perché i costi per riparare i danni prodotti da alluvioni, frane, inondazioni e terremoti sono molto superiori ai costi degli interventi in grado di prevenire gran parte di tali danni. È questa la ragione per cui il nostro Gruppo sostiene con forza l'emendamento 8.2 che, lo ripeto, mira al ripristino del Fondo regionale di protezione civile. Invitiamo pertanto i colleghi di maggioranza e il rappresentante del Governo a considerarlo con grande

senatori Bevilacqua e Gentile, che chiede la dotazione eccezionale di 80 milioni di euro per far fronte agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Calabria. Bevilacqua ha illustrato la drammaticità di questo ennesimo evento, che nasce anche e molto dall'inadeguatezza della prevenzione territoriale

di trovare le risorse che le imprese alluvionate stanno aspettando da anni,

Dico questo perché nel settembre del 2008, quindi pochi mesi fa, l'Unicredit - Mediocredito Centrale spa, che è il soggetto erogatore di queste risorse, ha comunicato che i fondi erano esauriti.

immediatamente trovare le risorse per queste aziende che, ripeto, hanno già sostenuto esborsi notevoli per rilocalizzarsi in aree non esondabili. Peraltro, la legge n.

prevedeva che quelle somme venissero destinate in modo prioritario proprio a questo tipo di interventi. Ho ritrovato

il rispetto della destinazione dei fondi previsti da tale normativa. Il ministro Giovanardi rispose che i proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale in questione erano pari a 418 milioni di euro nel 2002 e a 356 milioni di euro nel 2003. Ci sono quindi risorse importanti,

che l'emendamento 8.5, con cui proponiamo l'autorizzazione di spesa di 30 milioni per i territori colpiti dall'evento sismico che ha colpito le Province di Parma, Reggio Emilia e Modena, non sta nella logica della gara a chi chiede di più o nella richiesta di misure *una tantum*. Rappresenta infatti una esigenza minima e nasce da una stima rigorosa dei danni che viene rilevata dai tecnici degli enti locali, dai nuclei di valutazione regionale che stanno rigorosamente operando anche con modalità di controlli incrociati, secondo una scala di priorità dell'urgenza, del rischio degli interventi. Ebbene, i 30 milioni richiesti non coprono neppure il fabbisogno che riguarda la prima fascia di emergenza, cioè il pronto intervento, cioè il ripristino del danno immediato ovvero le condizioni minime di agibilità. quelle stime nelle tre Province sono ben oltre, come si è detto, 150 milioni di euro. Reggio Emilia da sola ha rilevato 50 milioni e questa stima non contiene la valutazione degli edifici privati. Questo per dare una dimensione. Com'è stato riconosciuto dal sottosegretario Bertolaso, gli enti locali hanno reagito con grande efficienza e prontezza. È un sistema di protezione civile che ha funzionato e non è la prima volta che il Sottosegretario lo porta ad esempio in tutto il Paese. Comuni, Province e Regione, in una azione integrata con il lavoro dei volontari, si sono assunti responsabilità dirette subito, senza attendere. Questi territori, signor Presidente, a fronte di tale sforzo si aspettano una risposta adeguata dal Governo. Il plauso fa piacere. A noi certamente fa piacere vedere riconosciuto un livello di qualità alto dei nostri governi locali. Ma questo deve diventare sostanza, deve diventare una risposta che corrisponda alla realtà dei fatti, nulla di più, perché quel sistema possa continuare ad essere davvero virtuoso, responsabile ed efficiente. Per questi motivi, il Gruppo sosterrà con forza l'emendamento 8.5.

apprezzo gli amici della Calabria e di altre Regioni che hanno avuto disgrazie negli scorsi mesi ed anni che reclamano giustizia. Spesso la classe dirigente, dopo i primi momenti, si dimentica delle tragedie che popoli e comunità locali attraversano. L'emendamento 8.7, signor Presidente, è sì per la mia Regione,

in cui - in questi giorni vengono ricordati dal processo di appello - sono morti 27 bambini, questi sì, come diceva il presidente Ciampi, lo voglio ricordare ancora una volta, per colpa di tutti noi, al di là delle responsabilità specifiche, perché certe misure di prevenzione non appartengono più alla cultura di questo popolo. Chiedo anche una verifica seria - lo chiedo agli amici della Lega sulle spese del terremoto del Molise, ma non potete lasciare per il primo anno nella storia delle calamità naturali e dei terremoti che non vi sia un euro in bilancio per continuare la ricostruzione. Devo informarvi, signor Presidente ed amici del Governo distratti, che il presidente Berlusconi, che dice di tenere tanto a cuore questa nostra Regione,

che vive ancora nelle capanne di legno tanto note. Questo nuovo modello Molise dov'è? Abbiamo un paese simbolo del terremoto che ha completato la ricostruzione, ma

sottoscritto alcune relazioni; credo che esageri pure quando chiede ancora 3 miliardi di euro, permettetemi però

per non bloccare la ricostruzione nel mio Molise e per intervenire in queste tragedie e calamità naturali di cui l'Italia è piena. Vi ringrazio.

i colleghi sanno, e se qualcuno non lo sa è bene ricordarlo, in Italia le compagnie che estraggono petrolio pagano la più bassa percentuale di *royalties*: soltanto il 7 per cento. Nel Regno Unito pagano il 50

anche se inalata in quote minime.

con l'emendamento 8.0.24 (testo 2), dopo un'ampia disamina della problematica che si è svolta in Commissione.

ad altro provvedimento, accogliendo in questa sede un ordine del giorno. Il parere è contrario sull'8.0.90/1

già ritirato i suoi emendamenti 8.0.203 e 8.0.204, in quanto abbiamo tutti convenuto che la materia dei dragaggi in aree portuali possa essere oggetto di specifico provvedimento e quindi di un'analisi più approfondita da parte sia delle Commissioni che dell'Aula.

senatore Belisario, la validità degli argomenti che ella ha svolto, sicuramente non è questa la sede più opportuna per entrare in temi di così delicata e sostanziale complessità.

ed altre. Perfino il paese del Presidente del Consiglio, Arcore, che è stato oggetto di una sospensiva di tre mesi di tributi e contributi, rientra in tale materia.

i dipendenti dello Stato che precedentemente erano stati esclusi e poi sono stati inseriti in quella categoria di dipendenti che potevano usufruire della sospensione.

dà la possibilità al Governo, tramite ordinanza, di regolamentare questi aspetti. Non deve accadere che un ente controllato dallo Stato possa mettere veramente nei guai intere popolazioni e soprattutto imprenditorie del Nord

Vi sono aspetti normativi sui quali confesso di non essere potuto entrare nel merito. Pertanto, mi rimetto al Governo.

ma l'INPS, a quanto ci viene segnalato, non ottempererebbe a questa linea, sì da richiedere la restituzione dei contributi non già in misura ridotta e scaglionata nel tempo ma in unica soluzione. PRESIDENTE. Scusi senatore, non so

che l'INPS in talune realtà venga a chiedere la restituzione dei contributi in unica soluzione e senza l'abbattimento che il Governo e il legislatore hanno stabilito. Se così è, molti privati e molte aziende si trovano in evidentissima e comprensibile difficoltà.

a zone e situazioni non destinatarie del beneficio stesso; questo non lo possiamo fare con un ordine del giorno e nella misura in cui questo ordine del giorno andasse oltre, è evidente che dal Governo verrebbe qualche fondata resistenza, ci piaccia o meno. Se, invece, la finalità è solo quella

‑ che non è acqua saponata, ma un documento del legislativo che è in qualche modo interpretativo della volontà legislativa e, quindi, efficace nel chiamare l'Esecutivo a intervenire sull'INPS. Se questo è lo spirito ‑ e lo è se il Governo e l'onorevole relatore verificano che la lettera non tradisce lo spirito, mi pare che possiamo diventare firmatari a più mani di questo documento che meritoriamente il senatore Astore ha presentato e approvarlo non come un rituale pezzo di carta, come spesso accade in questa e in altra Aula, ma come un documento interpretativo che dovrebbe finalmente esplicare la sua efficacia. Chiederei al relatore di precisare qualcosa in questo senso. Forse, possiamo fare qualcosa di concreto.

Sul resto, quello che posso garantire è un impegno del Governo a reperire ulteriori fondi, ma questo passa attraverso il ritiro degli emendamenti 8.200 e 8.201 e la contestuale presentazione di un ordine del giorno.

Sono presenti in tribuna l'ambasciatore del Marocco, Nabil Ben Abdallah, il primo consigliere e il ministro plenipotenziario, ai quali va il nostro saluto.

abbiano instaurato una nuova ipotesi di fallimento coatto, perché tutte le aziende che non avranno le risorse (il Governo si è opposto a questo) falliranno. Il Governo si assume una gravissima responsabilità.

già nel 2004 ci fosse stato un impegno da parte dell'allora ministro Giovanardi per dare una soluzione a questo problema che si trascina dal 1994. La proposta di inserire l'emendamento in questo decreto si rende necessaria sia per rispondere alla necessità d'intervenire con urgenza a favore di quasi 150 imprese che attendono da oltre un anno, a causa della carenza di cassa, la piena attuazione delle leggi citate, sia per proseguire l'opera di messa in sicurezza dei territori colpiti dai diversi eventi alluvionali che si sono registrati anche di recente in tutte le principali Regioni italiane, in particolare nella regione Piemonte. Nel provvedimento in questione viene preso a particolare riferimento l'articolo 3-*quinquies* della legge n. 17 del 2007, il quale ha prorogato i termini per accedere ai finanziamenti agevolati previsti dall'articolo 4-*quinquies* della legge n. 228 del 1997 e alle agevolazioni di cui all'articolo 1-*bis* della legge 19 ottobre 2004. Sulla base delle indicazioni fornite dagli enti gestori incaricati di esaminare le domande presentate dai soggetti beneficiari di cui alla citata legge n. 17 del 2007, è risultata, alla data del 19 settembre 2008, una carenza di cassa che, qualora non risolta, non solo non permetterebbe di proseguire anche in futuro la giù generale opera di messa in sicurezza e prevenzione nel territorio, ma vedrebbe lesi i diritti dei soggetti che hanno aderito nei primi due anni di attuazione alla legge citata. Risultano essere infatti 206 le imprese beneficiarie delle provvidenze che alla data della manifestata carenza di cassa si sono viste comunicare l'interruzione del servizio senza un'adeguata risposta relativamente alle prospettive di ripresa dell'erogazione dei contributi assegnati. Va inoltre rilevato che il mancato rifinanziamento della norma, oltre alla citata lesione procurata alle imprese, che con corposi investimenti hanno anticipato quanto loro dovuto dallo Stato ai sensi delle leggi in vigore, non consente il proseguimento delle opere per quanto attiene alle oltre 30.000 aziende potenzialmente interessate a beneficiare in futuro di tali provvedimenti. L'intervento normativo si pone l'obiettivo di colmare tale carenza mediante l'utilizzo delle risorse ad esso destinate ai sensi di quanto previsto dalla legge n. Infatti, al comma 1 dell'articolo 10 della citata legge n. 35 del 1995, è prevista la corresponsione di una cifra pari a 403 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2000, finalizzata a garantire la copertura finanziaria degli articoli 2 e 3 della suddetta legge. Tali risorse, generate ai sensi di un'addizionale sull'imposta di bollo, prevista ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 della legge n. 35 del 1995, concorrono alla copertura degli oneri di tale legge e sue successive modificazioni e integrazioni, ai sensi di quanto previsto dal primo capoverso del successivo comma 7. In altre parole, abbiamo creato le condizioni per avere una tassa di scopo, ma le risorse che continuiamo a raccogliere e che abbiamo raccolto in passato non le utilizziamo per l'obiettivo che ci eravamo posti. Per concludere, oltre ad evidenziare che si aggiunge anche la sottoscrizione del senatore Marcenaro, devo dire che mi stupisce veramente molto che il Governo abbia assunto questa posizione. posizione. Si può dire di voler tutelare il tessuto imprenditoriale del Nord; si può agire per tutelarlo sul serio: questa è un'occasione per agire e non per dire, ma mi sembra che la si voglia perdere con determinazione. Nonostante ciò a cui ormai ci stiamo abituando anche in quest'Aula, ritengo che la coerenza sia ancora un valore e ad essa faccio appello per questa votazione.

un ordine del giorno, che ho provveduto a consegnare entro il termine della seduta di ieri, che impegna il Governo stesso a valutare la possibilità di reperire il fabbisogno finanziario necessario agli interventi descritti in precedenza dalle risorse

Intendo anche evidenziare all'Aula, visto il tono polemico con il quale sono intervenuti gli altri colleghi piemontesi che rappresentano l'opposizione, che in questo particolare settore, fino a quando il collega

una grande fetta delle risorse che si erano venute a determinare in base a questo provvedimento specifico. Purtroppo, negli ultimi anni la Regione Piemonte ha dormito

si attardano in altre questioni, magari più ideologiche, come offrire la propria Regione per far morire la povera Eluana *(Commenti dai banchi del

oltre al problema della Calabria, il nostro Capogruppo si farà carico di segnalare, peraltro in conformità con l'ordine del giorno già accolto ieri sera dal Governo, le questioni relative all'argomento di cui stiamo parlando.

secondi per sottolineare che ha ragione il senatore Fluttero; pertanto, porteremo anche questa vertenza all'attenzione del Governo con l'impegno che l'ordine del giorno meriterà.

abbiamo seguito la logica della drammatizzazione mediatica. Si è fatto un patto di rigore, di responsabilità, per cui credo che bisogna dire sì o no a questo tipo di gestione della protezione civile e degli interventi in caso di danno. Questo è stato un evento esteso e molto profondo, che fa

proporrei di cassare il riferimento alle apposite ordinanze. Quindi il primo periodo del dispositivo dovrebbe essere formulato in termini più generici, come segue: «a garantire l'effettività della disposizione richiamata in premessa e ad adottare misure utili a chiarire che».

sostenere presso il Governo questo emendamento così importante, che per i distretti economici industriali della lavorazione del marmo riveste una grandissima importanza. I distretti in discussione sono dislocati in tutte le aree del Paese, principalmente nel territorio veneto, a Verona ed a Vicenza, in Toscana, nel distretto di Massa Carrara, ed in Sicilia, nel distretto di Trapani; tra estrazione e lavorazione del marmo una parte rilevante del PIL di quei territori è appunto sostenuta da questo segmento industriale. Tale comparto, quindi, è molto importante per la nostra economia, coinvolge molte società e moltissimi dipendenti. Solo in Veneto il distretto del marmo conta circa 500 aziende con più di 5.000 addetti, con una presenza forte ed organizzata. una grande opportunità che il Governo ha saputo cogliere per favorire in questo settore l'economia legata al reimpiego di tali materiali, con il conseguente mantenimento - e noi ci auguriamo anche l'aumento

mettiamo fine quindi ad un'impostazione che era stata data dal precedente ministro Pecoraro Scanio e che era fortemente penalizzante per queste aziende, grazie al Governo e grazie al lavoro della Commissione.

un'indagine molto puntuale e che quindi tutti i dati che sono stati indicati sono ben noti ai componenti della stessa, i quali hanno convenuto sul testo dell'emendamento. Quindi, non c'è nessuna primogenitura, ma un lavoro fatto costantemente e seriamente sull'argomento

semplicemente segnalare che all'emendamento 8.0.90 ed alla sua applicazione va riferito

servizi di depurazione connessi al più complesso servizio idrico, nei casi in cui i piani d'ambito e i gestori non siano in grado di fornire il servizio. La Commissione ‑ ripeto ‑ ha convenuto sul principio e ha una norma interpretativa del concetto di servizio di depurazione che ricomprende anche i costi dell'apprestamento delle infrastrutture necessarie a rendere il servizio, quindi la progettualità e gli investimenti relativi agli impianti di depurazione. Perciò, la legittima attesa dei cittadini al rimborso non verrà assolutamente negata; anzi, sarà confermata, ad eccezione delle quote di tariffa che afferiscono all'intero concetto di servizio di depurazione. precisi con decreto quali sono le voci che incidono su questo punto, tenendo presente che, comunque, tutti coloro che non sono allacciati al servizio di depurazione, perché non previsto dal piano (non per un'inefficienza del gestore, ma perché non sono previsti allacciamenti delle loro zone e delle loro utenze al servizio di depurazione), dovranno comunque corrispondere un

applicata, senza particolari traumi e impatti sulla finanza pubblica, da parte di tutti gli enti gestori per risolvere un problema che stava mettendo effettivamente in difficoltà numerose aziende di gestione ed enti locali.

di tale delicatezza che ritenevo opportuno informarne l'Aula, non solo in merito ai contenuti, ma anche alla genesi del provvedimento proposto. [DELLA

ad una decisione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Naturalmente la sentenza della Corte costituzionale, oltre a essere insindacabile, è anche condivisibile nel merito. È ovvio che tutti siamo d'accordo che chi ha pagato in modo improprio per un servizio non reso vada rimborsato. A noi ciò che preme è che nel dispositivo di applicazione di questa sentenza si tenga conto in maniera accurata di due

chi scarica le proprie acque reflue nei corpi ricettori senza che queste vengano depurate ha diritto sicuramente al rimborso di eventuali somme erogate per servizi non resi, ma è altrettanto indubbio che l'impatto ambientale dei suoi scarichi non depurati ha un costo, determina un danno. È chiaro che questo costo e questo danno debbono essere in qualche modo tenuti in considerazione nella definizione dei meccanismi di restituzione delle somme non dovute. Per questa ragione noi, riconoscendoci nei presupposti iscritti in questo emendamento, ci riserviamo però un giudizio finale nel momento in cui si potrà leggere la decisione concreta del Ministero dell'ambiente che definirà i meccanismi pratici di restituzione delle somme eventualmente non dovute. Questa è la ragione per cui su questo emendamento, di cui pure condividiamo l'impostazione e l'ispirazione, ci asterremo.

alla luce di due obiettivi: armonizzare la norma con la normativa europea e salvaguardare, nel contempo, la positiva esperienza sviluppatasi in questi anni in Italia nel campo della raccolta e dello smaltimento

saremmo dovuti abituare negli ultimi mesi, ma le continue pratiche di rinvio e la disapplicazione tramite proroga o deroga di disposizioni ambientali molto spesso di derivazione comunitaria non possono essere motivo di abitudine. La formulazione fumosa e contraddittoria della disciplina di transazione globale in materia di danno ambientale basterebbe da sé a motivare il voto contrario. In sintesi, vi è il rischio di "condono tombale" sull'inquinamento. Le norme sono frammentarie ed eterogenee; le modifiche aggiunte dal Senato sono peggiorative. Per

l'articolo 2, la risoluzione extragiudiziale del contenzioso, a proposito delle procedure di rimborso delle spese di bonifica e di ripristino delle aree contaminate, può comportare

Prego, senatore Pardi, alla transazione globale, bisogna osservare che mancano le cautele necessarie in ordine ai poteri di autorizzazione, controllo e vigilanza sulla facoltà di utilizzare il terreno a fini industriali e di azzerare con un pagamento le responsabilità accertate e quelle che potrebbero risultare a mano a mano che il danno ambientale viene ad emergere in tutta la sua gravità. Nel prosieguo si affida al solo Ministero la definizione di controlli. Si impone allo Stato di concordare con chi inquina perfino lo schema preliminare della proposta di accordo. In questa maniera, si apre la possibilità di un condono a pagamento per gravi episodi di inquinamento.

Mancano i requisiti di necessità ed urgenza: di fatto, si determina una delega in bianco al Ministero dell'ambiente a trattare con i grandi inquinatori e si crea un danno al principio comunitario di responsabilità e prevenzione ambientale. non si capisce il mancato riferimento ai lavoratori a tempo determinato di ISPRA e APAT per i quali dovrebbe, comunque, essere assicurata la possibilità di stabilizzazione già prevista dal Governo precedente. Agli articoli 5 e 6 siamo contrari per il continuo mancato adeguamento dell'Italia alle norme comunitarie sull'inquinamento delle falde idriche e rifiuti, siano essi rifiuti solidi urbani o rifiuti speciali. C'è poi uno specifico giudizio negativo sull'emendamento che modifica la composizione e la denominazione del Comitato per la vigilanza delle risorse idriche. Qui siamo di fronte a un espediente che determina una sorta di *spoil system*: si cambia la forma della nomina per nominare i nuovi membri, in omaggio appunto al nuovo meccanismo, sempre più diffuso, dello *spoil system*.

che impegna il Ministero dell'ambiente a promuovere la valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato. Non si capisce quale usato sia; non c'è specificazione. Sull'articolo 8 non sono state approvate le nostre proposte sull'abbattimento dell'inquinamento da idrogeno solforato su cui si sono intrattenuti vari emendamenti, cosa che ci viene, peraltro, richiesta dall'Organizzazione mondiale della sanità. Infine, non si è voluta rifinanziare l'operatività per il 2009 dei fondi regionali di protezione, azzerati dalla finanziaria 2009, né si è voluto trovare risorse aggiuntive per il proseguimento degli interventi relativi alle calamità naturali, illustrate dagli emendamenti dei colleghi (l'alluvione in Piemonte e il terremoto in Molise). L'insieme di tutti questi dinieghi e dell'aggravio di fattori di rischio ambientale e, soprattutto, l'apertura di una dimensione sostanzialmente discrezionale, che lascia all'autorità di Governo la possibilità di patteggiare, concordare e, in un certo senso, anche nascondere la relazione tra autorità politica, governo del territorio e risanamento delle zone inquinate, fa sì che l'opinione convinta del Gruppo dell'Italia dei Valori non possa che essere nettamente contraria.

dico subito che voterò a favore di questo decreto e che tutto il Gruppo che mi onoro di rappresentare lo farà convintamente. Si tratta di un decreto che rappresenta un primo tassello della rivoluzione ambientale che la potente 13a Commissione, di cui faccio parte, si è prefissata di compiere in questa legislatura. Sappiamo tutti che in materia di ambiente ci sono tante cose da fare, che tutti noi ne siamo responsabili e che tutti noi dovremmo essere promotori. Sono solito dire che l'ambiente è formato da tutti i colori dell'iride. La nostra è anche una responsabilità mondiale e vi spiego il perché: l'abate naturalista Antonio Stoppani, rosminiano, alla fine dell'800 definiva il Paese Italia il bel Paese. Con Stoppani nacquero i primi naturalisti e archeologi; fu anche un patriota: lottò nelle cinque giornate di fianco a Cattaneo e coniò la frase famosa «padroni a casa nostra».

provvedimento in esame si occupa di una molteplicità di questioni e molte altre sono state introdotte aggiuntivamente e continuamente fino alle ultime ore, fino alla discussione sugli ultimi articoli ancora questa mattina. Né vale l'idea che successivamente questi emendamenti siano stati ritirati:

in modo continuato e reiterato sono stati presentati alla nostra attenzione. Già l'uso continuativo, peraltro, della decretazione d'urgenza sulle più disparate materie è diventato il modo con cui il governo esautora il Parlamento delle competenze che gli sono proprie. Se ora aggiungiamo il metodo - questo metodo, peraltro già più volte seguito - utilizzato per questo decreto otteniamo un quadro sconfortante. Un decreto non può essere un provvedimento *omnibus* che il Governo utilizza a piacimento, incurante dei contributi parlamentari, ivi compresi quelli della sua maggioranza. Abbiamo assistito, infatti, nel dibattito su questo decreto ad una situazione veramente paradossale: tutti gli emendamenti, anche quelli significativi, presentati da esponenti della maggioranza sono stati ritirati altrimenti ci sarebbe stato il parere negativo. Non ho capito quale sia il problema vero che stia dietro un decreto come questo, su cui avremmo potuto lavorare seriamente in Commissione e probabilmente produrre risultati utili per l'intero Paese. Il testo è invece stato costruito e condotto al voto ignorando il contributo costruttivo e non ostruzionistico

La Commissione ha lavorato d'intesa su molti punti, come spesso accade, ma questo lavoro inspiegabilmente non è servito a molto. su molte delle questioni sono rimaste posizioni insanabili, proprio per il reiterato atteggiamento oppositivo del Governo. tuttavia sullo sfondo un elemento non trascurabile per il suo inesorabile ed ininterrotto ripetersi: l'assenza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del mare, sempre e continuativamente. L'assenza del Ministro è sistematica; non me ne voglia il sottosegretario Menia, che la minoranza ringrazia per la sua assiduità ai lavori ai lavori della Commissione sui vari argomenti che vengono affrontati. Ma il Ministro no, il Ministro non viene mai, non sappiamo che cosa pensi su argomenti importanti, pure trattati nel decreto in esame. Che cosa sarà del decreto‑legislativo n. 152? Quali parti il Ministro intende riformulare? A quali parti darà piena attuazione? Il regolamento qui citato, previsto dall'articolo 238 ed ormai in ritardo cronico, verrà mai emanato? Verrà emanato questo decreto? È vero che un emendamento del relatore ha cercato di rendere meno dirompente questo problema, ma il problema esiste. Sulle discariche dei rifiuti, quali politiche intende adottare il Ministro? Capisco che ci siano tipologie di rifiuti specifiche che rischierebbero di far saltare il sistema; ma perché non abbiamo ancora pensato almeno un piano per le tipologie che vengono considerate, in questo decreto, dove c'è un'ulteriore proroga sul mantenimento di talune discariche? Perché per altri Paesi europei ciò non è accaduto? Perché non ci preoccupiamo di dare piena attuazione alle direttive europee in materia ambientale? Perché oggi dobbiamo di nuovo approvare un articolo come l'articolo 6? Perché siamo fuori da qualunque capacità di previsione e di programmazione su materie su cui l'Europa ha già dato precise indicazioni? E ancora, vorrei chiedere sempre al Ministro a che punto sono la bonifica e la messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale. È vero, ci siamo scontrati sulla procedura, ma non c'è solo un problema di procedura sulle transazioni finali; non è la prima volta che il Partito Democratico lo chiede. Non solo non è venuta mai una risposta, ma addirittura in questo decreto viene proposta una frettolosa procedura transattiva che aprirà ulteriori contenziosi a catena. Condividiamo l'idea di velocizzare la chiusura di talune antiche - sottolineo antiche - questioni legate al danno ambientale nei siti di interesse nazionale, ma le modalità transattive qui previste non ci convincono, perché non tengono conto di una casistica complessa e varia e le conseguenze di questa mancata previsione saranno disastrose. *(Brusìo in Aula).* Colleghi, capisco che abbiamo tutti fretta di concludere

Signor Presidente, mi sembra che in quest'Aula, su indicazione del presidente Schifani

riferendomi ai provvedimenti in materia di protezione civile. Questi provvedimenti sono sempre emergenziali e transitori. Anche in questo decreto compare con chiarezza come i tagli imposti nei provvedimenti precedenti su problemi non certo secondari per il Paese, come il dissesto idrogeologico e la protezione dell'ambiente, ci impongano sempre di rincorrere i danni provocati da eventi naturali, siano essi il terremoto dell'Emilia Romagna o le recenti alluvioni in Calabria, con i cospicui danni che ne sono conseguiti. Siamo sempre in fase di rincorsa.

unico autore di tutto quanto abbiamo visto, non lo abbiamo mai saputo, né allora né in seguito, perché con il Ministro dell'ambiente non abbiamo mai potuto parlare e anche nel decreto in esame ne vediamo le conseguenze. Pochi e scarsi interventi sulle emergenze e sul resto si vedrà. Prendo atto delle dichiarazioni del senatore Gasparri sulla Calabria e poi sul Piemonte; speriamo che non siano un pannicello caldo per superare la mattina e arrivare velocemente alla conversione del decreto-legge senza creare problemi al Governo, perché è chiaro che su questi argomenti questa mattina un voto dell'Aula sarebbe stato sicuramente negativo per il Governo e contrario ai pareri che il Governo ha espresso in prima battuta su tutti gli emendamenti che riguardavano questi interventi; intanto, comunque, il dissesto continua. dissesto continua. Mi sono occupata, in questa mia dichiarazione, soprattutto del metodo, perché sul merito sono già intervenuta più volte. Mi chiedo però

reca scarsi segni di democrazia, secondo la quale se un organismo di controllo non è in scadenza e se ne vogliono sostituire i componenti, anche quando hanno ben operato e a prescindere dalla qualità dell'attività svolta, basta abolirlo e crearne un altro. Mi chiedo se questa e di serietà e come possiamo condividerlo. Qualcuno dirà che gli emendamenti alla fine non hanno avuto corso, ma l'idea c'è è stata e mi preoccupa, proprio perché dietro vi abbiamo visto questo metodo segnato da scarsa democrazia e da grande confusione. Certo, l'operazione non è andata a segno, ma lo spirito che l'ha condotta non ci piace, non lo condividiamo e speriamo che non abbia più a ripetersi. Pensate che l'emendamento 6.0.6, fatto presentare al relatore, sempre per dare una parvenza estetica a tutta la vicenda,

proponeva una Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche in luogo del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, anche in questo caso al solo fine di cambiarne i componenti; peraltro, la Commissione ha recentemente audito il Presidente del Comitato ed ha espresso plauso e parere favorevole sulla relazione che il Comitato ha reso alla Commissione. È democrazia questa? Che modo è di procedere? Che collaborazione si cerca? Qualcuno dirà che sono solo questioni di denominazione, ma non è così: i componenti di questi due organismi non erano né in scadenza, né avevano male operato, pertanto questo fatto, anche se rimasto solo nelle intenzioni, non ha alcuna giustificazione e ci preoccupa e giustifica ulteriormente il nostro voto negativo. Quello che noi censuriamo è il metodo. Non mi resta, a questo punto, che annunciare il convinto voto contrario del Gruppo del Partito Democratico al decreto in esame.

il Parlamento italiano ha disciplinato il tema del «chi inquina paga» con i poteri sostitutivi, con la nomina di commissari *ad acta*, con l'iscrizione di privilegi legali sopra le aree inquinate, con l'acquisizione coatta di abbiamo all'esame un provvedimento che declina il principio del «chi inquina, paga», prendendo in considerazione le ipotesi nelle quali l'inquinatore paga davvero, si rende disponibile a fare le bonifiche e a realizzare i piani di recupero e di messa in sicurezza. A questo caso, che purtroppo è stato tenuto in poca considerazione nel nostro ordinamento, si offre una risposta operativa convincente, che sbloccherà decine di bonifiche nel nostro Paese e che consentirà la ripresa di un settore che ha una forte ricaduta economica. Il principio del «chi inquina, paga» viene declinato senza pregiudizi ideologici e senza allarmismi, ma con criteri di efficacia delle norme che l'ordinamento realizza.

che abbiamo trovato in condizioni molto gravi, dal punto di vista non soltanto dell'ordine pubblico, ma anche - diciamo così - della convivenza pacifica, dell'igiene e della profilassi.

CIE. Auspichiamo che quanto prima, possibilmente entro la fine della settimana, una delegazione del Governo si rechi in quel luogo, perché da campo di identificazione ed espulsione sta diventando un vero e proprio campo di reclusione.